Signor Presidente, onorevoli senatori, il trasporto intermodale delle merci e, in particolare, quello connesso al settore della logistica e del trasporto ferroviario delle merci rappresenta un tassello rilevante per il perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione del settore del trasporto in linea con le politiche del *green deal* europeo. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) ha da sempre avuto un costante e proficuo confronto con le associazioni di categoria e con gli operatori del settore del trasporto ferroviario per la condivisione delle iniziative da intraprendere a tutela del comparto. Sono stati quindi promossi numerosi interventi a sostegno del settore, tra cui il contributo alle imprese ferroviarie per il pagamento del pedaggio ferroviario, il cosiddetto sconto pedaggio, con lo stanziamento di 100 milioni di euro per il periodo dal 2023 al 2027. Nel 2023 si è avuta una revisione e semplificazione delle procedure amministrative della verifica delle istanze presentate, che hanno ridotto sensibilmente i tempi per l'erogazione del contributo alle imprese. Sono state riconosciute altresì le contribuzioni alle imprese ferroviarie e agli spedizionieri conseguenti all'emergenza Covid, per un importo complessivo di circa 27 milioni di euro, di cui circa 25 imprese ferroviarie merci per il periodo 2020-2034 e circa 2 milioni per

In merito al ferrobonus*,* in seguito all'autorizzazione della Commissione europea, il MIT ha provveduto alla redazione di un nuovo regolamento che ha dovuto seguire l'ordinario *iter* procedurale. Il relativo decreto interministeriale MIT-MEF è stato definitivamente adottato il 30 agosto 2023. Lo scorso 6 ottobre il provvedimento è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* ed è entrato in vigore il successivo 21 ottobre. Nella stessa giornata è stato pubblicato il decreto direttoriale recante le istruzioni operative per la presentazione delle domande di accesso al contributo per le annualità 2023-2024, al fine di garantire la tempestiva erogazione delle risorse alle imprese operanti nel settore del trasporto intermodale e trasbordato, da e verso nodi logistici e interporti italiani. Per le risorse relative all'esercizio 2023, le stesse saranno erogate in forma di acconto sulla base di stime effettuate sullo storico del traffico "ferrobonus". Tale meccanismo ha consentito l'utilizzo a favore dei beneficiari del ferrobonus di tutte le risorse statali allocate per l'attuazione della misura incentivante per il 2023. La risposta all'interrogazione mi consente di informare l'Assemblea sugli esiti dell'istruttoria documentale che si è conclusa il 18 dicembre 2023. Sono state presentate 82 domande, di cui 81 ammissibili. Il successivo 19 dicembre il MIT ha emesso il relativo decreto d'impegno registrato dall'Ufficio centrale di bilancio il 15 gennaio scorso, per un importo complessivo di 22 milioni di euro per l'annualità 2023. Tutta la documentazione è reperibile sul sito istituzionale del MIT. Al momento sono in corso le operazioni propedeutiche per la liquidazione degli ordini di pagamento alle imprese ammesse al contributo. Infine, per quanto attiene agli investimenti, il soggetto gestore Rete ferroviaria italiana ha rappresentato che il piano industriale 2023-2032 prevede significativi interventi per la rete per i servizi merci, tra i quali segnalo: l'*upgrade* prestazionale del corridoio merci con gli adeguamenti prestazionali agli *standard* per la rete «core» TEN-T al 2030; il rafforzamento del primo-ultimo miglio per migliorare l'accessibilità della rete e l'integrazione con le altre modalità con il collegamento tra l'infrastruttura ferroviaria nazionale con porti e terminali. Al 2032 saranno realizzati tre nuovi collegamenti ferroviari e potenziati nove collegamenti già esistenti con porti e dodici collegamenti con terminali terrestri; l'ottimizzazione dell'offerta di capacità per i servizi merci e specializzazione degli itinerari ed infine sviluppo di servizi di logistica intermodale per la digitalizzazione dei processi, attraverso la realizzazione di un sistema informativo, il progetto "*Easy rail freight"*, ad uso di tutti gli attori della catena logistica.

In più, ci sarebbe il fatto che - anche a dispetto del suo nome - le politiche a sostegno del ferro di questo Governo sono incerte, deboli e probabilmente anche figlie della non convinzione intorno al *green deal*, che pure lei ha citato. La parola principale, però, è appunto "tempo". Dopo oltre sei mesi dalla presentazione dell'interrogazione, in particolare per l'impegno del senatore Basso, che ringrazio, siamo riusciti oggi ad ottenere una risposta dal Governo. Non possiamo ritenerci soddisfatti, prima ancora di entrare nel merito della questione trattante, in quanto questo tempo trascorso non è una variabile indipendente rispetto alla rilevanza dei temi in questione. Per il settore di cui stiamo discutendo, come e più di tanti altri comparti dell'economia del Paese, il tempo è una componente fondamentale, che può fare la differenza nell'avanzamento di innovazione e sviluppo del settore. Lo è, ovviamente a parti inverse, in negativo, anche il tempo perso. del cosiddetto ferrobonus non se ne è perso poco, purtroppo. Oggi, tramite lei, il Governo viene a dire davanti a quest'Assemblea, che ha fatto, che si è impegnato, che ha messo in campo dei provvedimenti, di cui prendiamo atto. Non si può, però, né sottovalutare né tacere che la vicenda oggetto di risposta del Governo è motivo di dibattito pubblico purtroppo da tempo. È trascorso quasi un anno da quando le associazioni italiane del trasporto ferroviario, Assoferr, Fermerci e FerCargo, si rivolgevano al ministro Salvini per avere notizie certe rispetto alle ripetute e svariate promesse sulla effettiva messa a terra dei benefici di legge. I rappresentanti delle associazioni espressero forte preoccupazione per il grave ritardo nell'attuazione di una misura che rappresenta una forma di sostegno imprescindibile per l'intera filiera intermodale del trasporto ferroviario delle merci, a condizione che venga corrisposta annualmente, in assoluta continuità e senza ritardi. Queste sono le loro parole, a me pare abbastanza inequivocabili. Una preoccupazione, quella espressa dalle associazioni di categoria, suffragata dal fatto che la misura del ferrobonus, già finanziata dal Governo Draghi fino al 2026, nonché approvata dalla Commissione europea fino al 2027, non ha trovato per lungo tempo nel Ministero dei trasporti un interlocutore attento e sensibile. pur sapendo che un ritardo nell'attuazione della misura avrebbe impedito la necessaria continuità con le annualità pregresse, determinando gravi ed evidenti conseguenze, in termini economici e occupazionali, per i settori produttivi nazionali del *cluster* ferroviario. Ma non sono le uniche conseguenze negative determinate dalla mancata tempestività delle scelte del Governo. Ciò che maggiormente emerge è l'assenza di una strategia in materia di transizione energetica o, per meglio dire, ciò che emerge ancora una volta è una conferma dell'assenza di visione su questo tema. È indubbio, è indiscutibile, che aver perso mesi rispetto alla possibilità di mettere in campo tempestive misure di sostegno ha significato perdere occasioni fondamentali nella possibilità di accelerare sulla transizione dalla gomma al ferro: una sfida cruciale per il sistema Paese, senza la quale non saremo in grado di raggiungere *standard* di sviluppo e sostenibilità moderni. L'obiettivo del trasporto combinato ferro-gomma merita di essere perseguito e sostenuto, con un'avveduta azione di Governo che concentri risorse vere, per rendere strutturale la misura del ferrobonus, se non altro perché, tra l'altro, incentivare l'intermodalità significa anche attivare strumenti per lenire la speculazione energetica e rendere il sistema Paese meno esposto. Per farlo bisogna fare l'opposto, mi sia consentito anche un cenno territoriale, di ciò che Fratelli d'Italia attua al governo del Paese e delle Regioni. Posso portare, con cognizione di causa, l'esempio della mia Regione, dove, dopo cinque anni di governo a trazione Fratelli d'Italia, il tema dell'intermodalità è derubricato a questione minore. Basti pensare che il Governatore, uomo di fiducia del presidente Meloni, non ha battuto ciglio nei confronti del Governo centrale, pur subendo un taglio di un miliardo e mezzo di euro nell'ambito della rimodulazione del PNRR per le risorse destinate alla ferrovia Roma-Pescara. un tracciato fondamentale per lo sviluppo del Centro Italia all'interno della trasversale Barcellona-Ploce. Una vicenda territoriale, ma eloquente, che chiarisce in modo adamantino quale sia il livello di carenza programmatoria e di visione che esprimono le forze politiche che governano il Paese. conclusione, è che questa interrogazione possa essere una volta ancora un richiamo al Governo a cambiare rapidamente strategie e priorità, ponendo in testa alle urgenze una strategia di transizione energetica che individui nel trasporto

è stata ricostituita l'alta commissione di cui all'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la valutazione delle proposte di rimodulazione relative al Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (Pinqua) nonché delle proposte progettuali riguardanti il programma sperimentale Dateci spazio. Dalla ricostituzione di detta commissione, a partire dal 2 maggio 2023, si sono tenute sedici sedute, l'ultima delle quali lo scorso 23 gennaio. La risposta all'interrogazione mi consente di informare l'Assemblea sugli esiti dei lavori della commissione e fornire un aggiornamento sul numero di richieste valutate e dei prossimi incontri. Ad oggi, sono state valutate positivamente 101 richieste di rimodulazione dei progetti inerenti al Pinqua. Soltanto per due è stato espresso un parere sfavorevole. La prossima riunione è stata già fissata per il prossimo 26 febbraio. Le rimodulazioni delle proposte oggetto di valutazione da parte dell'alta commissione intervenute dal 2 maggio 2023 ad oggi non hanno comportato criticità tali da mettere in discussione il relativo finanziamento concesso e sono tutte in linea con il rispetto delle tempistiche del PNRR e del programma in particolare. Per completezza di informazione, si comunica che per il programma Dateci spazio sono stati presentati 12 progetti, di cui 11 ammessi a finanziamento.

per le attività che ha intrapreso e che hanno in qualche maniera posto fine a una situazione paradossale. l'alta commissione per la valutazione dei progetti Pinqua è rimasta in qualche maniera bloccata per molto tempo perché due dei membri che ne facevano parte erano stati posti in quiescenza e non erano stati sostituiti. Però, signor Sottosegretario,

Il problema è che stanno partendo dei lavori, so che anche questo sta succedendo nella mia città, però è iniziata una corsa contro il tempo perché questi devono essere ultimati entro marzo 2026. ovviamente al Governo di non abbassare mai la guardia e monitorare sia la qualità che la concreta esecuzione di questi lavori. Posso dire che nella mia città

porre particolare attenzione a quei territori perché altrimenti rischiamo di avere tanti cantieri aperti, ma quasi nessuno di essi riuscirà poi a portare a termine i lavori.

Abbiamo parlato tempo fa del decreto-legge Caivano, a proposito del quale abbiamo visto che la politica di questo Governo si era preoccupata un po' troppo di dare una risposta

l'autonomia differenziata e la cosa che più mi è dispiaciuta di questo provvedimento è che in Commissione avevamo fatto di tutto per segnalare la necessità di una perequazione infrastrutturale, che richiedeva sì degli investimenti, ma che avrebbe creato le stesse condizioni e le stesse opportunità di sviluppo in ogni angolo d'Italia. I progetti Pinqua riguarderanno tutto il territorio nazionale. Quello che avete fatto con l'autonomia differenziata sta togliendo la speranza a quei territori che hanno gravi carenze infrastrutturali che impediscono alle imprese di investire, perché nessuno mai penserà di investire dove non ci sono aeroporti, autostrade e collegamenti sufficienti. Quindi, rivolgerei un ulteriore appello per un secondo ravvedimento operoso: fate in modo che questo *gap* si possa colmare, perché tutta l'Europa si sta muovendo in quella direzione. Le politiche di coesione europea vogliono eliminare anche i *gap* infrastrutturali. Quello che hanno fatto altri Paesi come la Spagna nell'Andalusia e nelle Isole Canarie, quello che ha fatto l'Irlanda nelle aree interne, quello che ha fatto il Portogallo devono essere degli esempi per farci capire che anche noi abbiamo la possibilità di far crescere l'Italia e di renderla di nuovo unita.

Anche le previsioni per il 2023 sono più che positive, come dimostrano i dati dell'*export* resi noti dall'Associazione nazionale fabbricanti di articoli ottici nei primi mesi del 2023, che registrano una variazione percentuale del 16,7 per cento in più rispetto ai dati del 2022. Secondo i più recenti dati forniti dall'agenzia ICE, la metà dei maggiori produttori su licenza sono situati in Italia e coprono il 50 per cento della produzione mondiale di licenze. Inoltre, il 90 per cento della produzione dell'occhialeria italiana è destinata ai mercati esteri. L'area di riferimento per le esportazioni italiane di occhiali da sole e montature è rappresentata anche nel 2022 da Stati Uniti e dall'Europa (in particolare Francia, Germania e Regno Unito). Orbene, al fine di tutelare il settore in parola,

e delle industrie italiane. In particolare, con l'approvazione della legge sul *made in Italy* dello scorso 27 dicembre sono state introdotte diverse novità per sostenere la produttività delle industrie italiane, ponendo una forte attenzione sulla tutela del *made in Italy*, al fine di difenderlo da azioni scorrette sul mercato che ne possano compromettere l'intrinseco valore riconosciuto in tutto il mondo. *In primis*, tengo a sottolineare che tale legge ha previsto l'istituzione del Fondo nazionale del *made in Italy*, cosiddetto fondo sovrano, partecipato dal MEF, aperto alla partecipazione di fondi di investimento e ad altri soggetti. La *mission* del fondo è quella di consentire maggiori investimenti nelle filiere produttive italiane, con l'obiettivo di rafforzare l'industria Paese, in coerenza con gli obiettivi di politica industriale ed economica prefissati. È stato altresì istituito il contrassegno ufficiale del *made in Italy*, che attesta l'origine italiana delle merci che le imprese producono sul territorio nazionale, al fine di tutelare e promuovere la proprietà intellettuale e commerciale di beni di origine italiana, attivando così un efficace contrasto alla falsificazione (come sapete, c'è il problema dell'*italian* *sounding*). Inoltre, è stato previsto un potenziamento delle norme in materia di lotta alla contraffazione e *italian sounding*. In tale direzione è stato previsto altresì che le fasi di lavorazione dei prodotti vengano certificate attraverso le *blockchain* e la creazione di un catalogo nazionale trasparente ed accessibile, per il censimento delle soluzioni conformi alla normativa in vigore sulla tracciabilità delle filiere, ai fini informativi del consumatore. Si è poi ritenuto necessario un intervento normativo sulle indicazioni geografiche, demandando alle Regioni la possibilità di effettuare una ricognizione delle produzioni artigianali industriali, le quali reputazioni sono strettamente connesse al territorio locale. Si ricorda infine l'istituzione del fondo speciale per la transizione verde e digitale della moda, che stanzia 5 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni di euro per il 2024. L'obiettivo è quello di sostenere il settore tessile della moda e degli accessori, con riferimento alla promozione e al potenziamento degli investimenti funzionali ad assicurare una transizione ecologica e digitale. La legge sul *made in Italy*, dunque, rientra nell'ambito di un'ampia strategia di questo Governo, che punta proprio a mettere le aziende italiane in condizione di competere sul mercato globale, da un lato, e di essere garantite da forme aggressive di concorrenza sleale, dall'altro.

Con particolare soddisfazione vediamo che questo Governo persegue e anzi intensifica la lotta contro la contraffazione, contro le scorrettezze e contro tutte le possibili manovre elusive delle norme esistenti.

Sotto questo profilo, infatti, la norma sul *made in Italy* sottolinea un particolare veramente importante, l'informazione del consumatore, perché *made in Italy* può essere tanto, ma occorre sapere bene cosa si intende quando si parla di produzione italiana. quindi avere una filiera trasparente, conoscere quel prodotto e dare la possibilità al consumatore di scegliere un prodotto italiano, perché prodotto in Italia, sapendo che è stato fatto con il *design* italiano, con la creatività italiana e con la produzione italiana. Ringrazio ancora il Governo e il sottosegretario Bitonci.

Signor Presidente, ringrazio il senatore Martella e i colleghi interroganti. Con riferimento all'interrogazione in parola, tengo a precisare che senz'altro per l'attuale Governo il gruppo Pirelli, storica società italiana, è di rilevanza strategica per l'interesse nazionale per le sue tecnologie all'avanguardia, la sua capacità di innovazione e la qualità dei suoi prodotti. Pertanto, lo scorso giugno si è ritenuto opportuno esercitare tempestivamente i poteri speciali richiamati dal senatore interrogante sull'operazione oggetto di notifica da parte di China National Tire & Rubber Corporation, riguardante il patto parasociale sulla *governance* della società Pirelli SpA. In particolare, rappresento che l'operazione notificata ha riguardato un progetto inerente nuove tecnologie sviluppate dal gruppo, le quali consentono ai cosiddetti sensori *cyber* impiantati all'interno dei pneumatici, di acquisire in tempo reale un'ampia gamma di dati, tra cui i modelli di traffico e di comunicazione terrestre, lo stato attuale di infrastrutture e la geolocalizzazione dei veicoli. Per questo motivo, i competenti uffici del Ministero, unitamente al gruppo di coordinamento della *golden power* istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, hanno ritenuto opportuno e necessario esercitare i poteri speciali con l'imposizione di diverse prescrizioni, non solo nei confronti della controllante cinese, ma anche nei confronti della stessa Pirelli SpA. Il fine è quello di preservare l'indipendenza industriale di Pirelli e del suo *management* nei processi decisionali, garantire la sicurezza delle procedure interne e tutelare la riservatezza dei dati raccolti attraverso le tecnologie sviluppate da Pirelli e il valore del suo *know-how*. La decisione del Governo, oltre a riconfermare alcuni impegni precedentemente assunti dall'investitore straniero, costituisce uno specifico strumento giuridico che consente a Pirelli di adottare idonee iniziative, soprattutto di carattere organizzativo, finalizzate a una maggiore indipendenza gestionale degli attivi riconosciuti strategici.

Tale monitoraggio avviene in accordo con la società, la quale è tenuta a inviare all'amministrazione una relazione redatta dal collegio sindacale, con la quale sono comunicate le misure adottate in osservanza delle determinazioni assunte con il DPCM e qualsiasi altra misura societaria o aziendale rilevante in rapporto alle stesse.

In effetti, il Governo ha attivato i poteri speciali della *golden power* per prevedere alcune prescrizioni, come lei ha ricordato, da rispettare nei confronti del socio privato che detiene la maggioranza azionaria in Pirelli e non solo nei confronti del socio privato, ma anche attivando quelle procedure di monitoraggio a cui ha fatto riferimento. Noi abbiamo esercitato la nostra funzione parlamentare di vigilanza e di controllo nei confronti del Governo, perché riteniamo che mantenere in Italia il controllo azionario e manageriale del gruppo Pirelli rappresenti, per storia, dimensione e tecnologie avanzate, un risultato importante per una delle più importanti aziende del nostro Paese e per uno dei *brand* più conosciuti al mondo. Devo dire però che si tratta di uno dei rari casi in cui il Governo ha tenuto conto delle nostre indicazioni. In questo caso è avvenuto nel mese di giugno, ma sono tanti gli altri casi di cui dovremmo parlare e su cui ci dovremmo attivare con efficaci azioni sia di carattere parlamentare che di carattere governativo. Stiamo vivendo infatti una vera e propria stagione di riorganizzazione dell'economia globale: sono trasformazioni che mai come oggi toccano l'industria. Certo, le implicazioni per tutta l'economia, a cominciare da quella dei servizi avanzati, sono enormi, ma è proprio l'industria ad essere al centro ed è proprio sull'industria che si gioca la partita del futuro. Non c'è dubbio che dovremmo puntare a digitalizzazione, sostenibilità e autonomia strategica e che questi siano gli obiettivi italiani ed europei verso i quali tutti dovremmo sentirci impegnati per mantenere la competitività del nostro Paese, ma rispetto a questi obiettivi Paese, ma rispetto a questi obiettivi non troviamo risposte da parte del Governo. Anzi, il Governo non ci appare capace di indicare delle vere politiche industriali, di sostenere davvero le imprese del nostro Paese e di aiutare veramente le filiere di carattere strategico, di garantire davvero un approvvigionamento sostenibile di materie prime. Non ci pare capace di incentivare il ritorno a casa di produzioni o di garantire una distribuzione territoriale che possa tenere insieme la competitività con la coesione sociale. Dico sociale. Dico tutte queste cose perché Pirelli è solo uno dei tanti tasselli di preoccupazione rispetto a quest'assenza di politiche industriali e di regia da parte del Governo. Quanto sta accadendo per l'ex Ilva è sotto gli occhi di tutti, visto che l'Italia sta correndo il rischio di perdere l'acciaio e sappiamo quanto questo possa voler rappresentare per un Paese che ancora si definisce industrializzato. stesso discorso vale per Stellantis: leggiamo le polemiche anche di queste ore, ma c'è un'enorme incertezza sul destino degli stabilimenti presenti in Italia e in generale su tutto il settore dell'*automotive*, in difficoltà nel passaggio dal termico dal termico all'elettrico. Accenno inoltre per ragioni di tempo alla questione della rete TIM, un assetto strategico infrastrutturale in uno degli ambiti più complessi del sistema economico del nostro Paese. Accenno poi davvero brevemente agli investimenti sfumati di Intel per tutte le questioni relative a *chip* e *microchip* o ancora alla trattativa tra Ita e Alitalia. Insomma, sono tutte questioni rispetto alle quali ci vorrebbe una regia pubblica delle politiche industriali, un intervento da affrontare come una priorità, non per dirigismo, ma come difesa degli interessi nazionali, come difesa degli *asset* industriali. Per concludere, mi riferisco infine ai 20 miliardi di privatizzazioni di cui avete parlato; 20 miliardi che non si capisce a che cosa servano, se per fare cassa o quale sia il disegno industriale che anima un progetto di tutto quel genere. Noi su questo punto le diamo atto della risposta, ma su tutte le altre cose che ho detto continueremo a svolgere la nostra azione, perché pensiamo che in Italia ci debbano essere delle politiche industriali e perché riteniamo che l'Italia debba continuare ad essere un Paese industrializzato.

acquisito nell'ambito dei piani di reindustrializzazione dell'area ex Whirlpool di Teverola. Il 26 aprile 2018 sono state concesse agevolazioni per complessivi 36,6 milioni a valere su risorse rese disponibili dal Ministero e dalla Regione Campania con l'accordo di sviluppo sottoscritto il 23 agosto 2017. Tale accordo prevede un incremento occupazionale di 85 unità lavorative per anno, di cui almeno 75 esuberi ex Indesit (gruppo Whirlpool); questi ultimi, da quanto riferito dal soggetto gestore Invitalia, risultano assunti già dall'esercizio 2020. Invitalia ha altresì comunicato che il progetto di investimento produttivo si è in parte concluso nel 2019 e che le agevolazioni sono state integralmente erogate. In particolare, si rappresenta che il progetto di ricerca, sviluppo e innovazione si è concluso limitatamente alla parte ricerca industriale, mentre è ancora in corso la parte per lo sviluppo sperimentale. È stata quindi richiesta una proroga per l'ultimazione del progetto di ricerca, sviluppo e innovazione fino al 31 dicembre 2023. 2023. Ciò in quanto, come comunicato dalla società, le attività da completare relative alla componente di sviluppo sperimentale si riferiscono all'installazione e messa in funzione di un ultimo macchinario (*mixer*), necessario per il completamento di uno dei due impianti pilota oggetto del progetto di ricerca e sviluppo. Si evidenzia, tuttavia, che la proroga non è stata ancora perfezionata, alla luce di alcuni accertamenti da parte del soggetto gestore. All'esito dell'istruttoria effettuata con i competenti uffici, risulterebbe che l'impresa abbia chiesto un incontro con Invitalia per valutare una rimodulazione del progetto di sviluppo sperimentale, per il quale resta da completare un ultimo impianto con costi previsti pari a 8 milioni di euro. In conclusione, si conferma che il Mimit continuerà a monitorare la situazione del sito produttivo in parola e il rispetto degli impegni presi. L'eventuale convocazione di un nuovo tavolo potrà essere considerata anche in esito alle valutazioni del soggetto gestore sul progetto in corso.

al contratto di sviluppo per la reindustrializzazione delle presenze ex Whirpool-Indesit in quel territorio. Il quadro che ne emerge è comunque, anche nella sua risposta, di un grave ritardo rispetto agli impegni che erano stati assunti, che - vorrei ricordarlo

2. Credo che lei abbia presente di che zona del Paese stiamo parlando: una provincia che definisce se stessa terra di lavoro, ma che è oggi costellata pressoché esclusivamente da aziende e aree di crisi dove si fanno grandi progetti, si promettono grandi soluzioni e poi iniziano inenarrabili e lunghissime vertenze che ogni volta vedono il modificarsi dei piani e dei progetti e nessuna delle risposte occupazionali che sarebbero necessarie. Questa è la ragione per cui mi permetto di chiedere che l'ex Ministero dello sviluppo economico, ora Ministero delle imprese e del *made in Italy*, convochi comunque un tavolo che affronti l'insieme di quell'area di crisi, cioè da un lato lo stabilimento per il litio e dall'altro lo stabilimento cosiddetto Teverola 2, di cui non si hanno non si hanno notizie (non riescono ad averle neanche le organizzazioni sindacali sul posto). Penso, infatti, che se è stato utile e necessario costruire le aree di contratto di sviluppo, costruire le aree di crisi, mettere a disposizione risorse, in questo caso del Fondo sociale e della Regione al fine di attuare la reindustrializzazione, ci sia un dovere collettivo che è quello che quelle risorse vadano a buon fine e si traducano effettivamente nella definizione di posti di lavoro. Credo anche, parlando di quel territorio e dello straordinario bisogno del Mezzogiorno di avere investimenti e di qualificazione, che siccome i progetti che riguardavano quest'area erano esattamente progetti che guardavano alla trasformazione - mi all'innovazione e ai settori connessi all'*automotive,* di cui parliamo tanto, ma di cui poi poco si traduce in termini di effettiva transizione e di innovazione industriale - questo abbia un interesse per il territorio, ma abbia anche un interesse di ordine generale. Da questo punto di vista, anche in accordo con le cose che ha appena detto il senatore Martella sulla politica industriale di questo Paese, vorrei sottolineare che c'è bisogno di politiche industriali per il Paese, ma c'è soprattutto bisogno di politiche industriali per il Mezzogiorno. Nel territorio del casertano, tutte le multinazionali se ne stanno andando, lasciando processi di reindustrializzazione senza fine, senza conclusione e senza soluzione e credo che questo non possa avvenire limitandosi all'attività delle amministrazioni locali o nella ricerca, come purtroppo siamo costretti a fare, di ammortizzatori per proteggere il reddito di quei lavoratori senza che ci sia alcuna speranza. Il mio augurio, quindi, è che il Ministero decida rapidamente di aprire un un tavolo di confronto per avere il quadro effettivo sia su Teverola 1 che su Teverola 2.

risponderanno il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro della salute. Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso.

Fratin per la sua disponibilità. Noi sappiamo che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da lei guidato, ha avviato una consultazione pubblica sullo schema di decreto che serve a definire gli incentivi tariffari per la produzione di idrogeno a basse emissioni di carbonio. Lei stesso ha evidenziato come il Governo punti molto sul vettore idrogeno e come sia necessario compiere un altro passo avanti per completare il il quadro di misure regolatorie e incentivanti già attivate in ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si tratta del principale provvedimento per stimolare gli investimenti nei settori industriali che risultano oggi più inquinanti e più difficili da riconvertire ed è necessario anche per l'utilizzo nei trasporti, con l'obiettivo, appunto di introdurre l'impiego di idrogeno, vettore energetico fondamentale per la decarbonizzazione. Le Regioni e le Province autonome possono, quindi, manifestare il proprio interesse per la selezione di progetti per la realizzazione di siti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse, da finanziare con le risorse del PNRR. Un testo importante, perché intende riconoscere agevolazioni sia ai produttori di idrogeno rinnovabile mediante processo elettrolitico, che di bioidrogeno, ottenuto da fonti quali bioliquidi, biomasse solide, biogas e biometano. Fatte queste premesse, gentile Ministro, le chiediamo quale sia il cronoprogramma previsto per la produzione di idrogeno, quali siano gli incentivi che verranno previsti per attivare queste misure, quali siano le ricadute positive concrete sull'ambiente attraverso la riduzione dell'intensità di carbonio e, quindi, il minore inquinamento, ma soprattutto

sottolineo che, in linea con la strategia europea sul tema, verranno implementate iniziative volte alla creazione di una filiera industriale dell'idrogeno, anche attraverso l'efficientamento delle prestazioni degli elettrolizzatori, al fine di garantire l'uso di tale fonte nell'industria cosiddetta *hard to abate* e nel settore dei trasporti, naturalmente con evidenti benefici in termini di competitività delle imprese italiane che si riverbereranno anche sui costi dei consumatori finali. Sulla base di REPower EU, l'obiettivo è produrre 10 milioni di tonnellate e importare 10 milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile nell'ambito dell'Unione europea entro il 2030, facendo divenire l'Italia uno dei principali *hub* europei (pensate che per le importazioni dovrà venire gran parte dal Sud) attraverso lo sviluppo del corridoio per l'idrogeno, in piena attuazione del Piano Mattei. Nello scenario di Polis 2030, delineato nell'aggiornamento del Piano nazionale integrato energia e clima, la quota di idrogeno rispetto al totale dell'idrogeno usato dell'industria salirà dal 3 al 42 per cento, in linea con gli obiettivi europei. La misura posta in consultazione ha come *target* un contingente di produzione di idrogeno rinnovabile al 2027 pari a 250.000 tonnellate e di 50.000 tonnellate di bioidrogeno. Il meccanismo incentivante ipotizza in questo momento, all'esito poi delle procedure competitive ad asta, un contributo in conto esercizio per la durata di dieci anni. Tale agevolazione è pari al maggior costo connesso alla produzione di idrogeno rispetto ad un combustibile convenzionale, con un valore massimo, in relazione alla tipologia dell'idrogeno prodotto, e alla dimensione dell'impianto variabile tra i tre e i cinque euro al chilogrammo. Sotto il profilo ambientale l'idrogeno deve soddisfare il requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita con una percentuale del 73,4 per cento rispetto a un combustibile fossile di riferimento; vale a dire che l'idrogeno promosso con la misura deve produrre meno di meno di tre tonnellate di CO2 per ogni tonnellata di idrogeno. La misura pertanto si pone come uno degli strumenti principali della strategia nazionale dell'idrogeno per la cui definizione è istituito al Ministero il tavolo tecnico. Quest'ultimo avrà il compito di individuare le linee di indirizzo sulla base del quadro regolatorio che si sta definendo in ambito europeo sulla *governance* e pianificazione infrastrutturale del settore idrogeno. Ricordo che l'Italia ha già investito sull'idrogeno, tra PNRR e fondi nazionali, oltre 3,5 miliardi. L'idrogeno è l'elemento più diffuso al mondo, ma è anche inodore e incolore e quindi la questione va trattata con molta cautela.

Ci convince anche la volontà di affrontare le tematiche dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili in contesti difficili, come quelli delle aree industriali. È importante anche rilevare la volontà di coinvolgere i territori, come le Regioni e le Province autonome, nella gestione di questi processi di produzione di energia in energia pulita. Da ultimo apprezziamo la sua volontà di non sprecare un centesimo dei fondi europei che abbiamo a disposizione, impiegando quindi i Il Parlamento, secondo me, non può che essere orgoglioso di questo suo lavoro, che è svolto davvero con grande responsabilità per il benessere di tutto il Paese e dei cittadini italiani.

è stato istituito anche un nuovo percorso di formazione, un percorso liceale del *made in Italy*, a partire dall'anno scolastico 2024-2025.

futuro di questo liceo del *made in Italy* e soprattutto sul destino dei licei economico-sociali. A quanto si apprende dal sito del Ministero, sono solo i licei ad indirizzo *made in Italy* finora approvati sul territorio nazionale. Un risultato che a noi pare deludente e che probabilmente è anche il frutto di una scarsa conoscenza del fatto che le scuole sono preoccupate,

con particolare riferimento ai licei economico-sociali e quale sarà il destino dei licei economico-sociali in mancanza di attivazione dei percorsi del liceo del *made in Italy*.

abbiamo ereditato un sistema formativo che evidenzia una profonda incapacità di formare proprio quelle professionalità maggiormente richieste dal nostro sistema produttivo. La gravità del ritardo accumulato in passato ha imposto la necessità di un'azione rapida da parte del Governo, che ha messo in campo più strumenti per aggredire da subito il *mismatch*, il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, che, come noto, tocca in alcuni casi punte anche del 60 per cento. Alle famiglie è stata offerta dunque maggiore possibilità di scelta per i propri figli, grazie all'introduzione di due novità, ossia la filiera tecnologica professionale ed il liceo del *made in Italy*. Due novità che, nella loro differente specificità, sono complementari ed integrano l'offerta complessiva. La scelta dell'attivazione di tali innovazioni è stata riservata, per mio fermo intendimento, alla piena libertà delle istituzioni scolastiche, che si sono espresse attraverso la deliberazione degli organi collegiali che ne rappresentano la comunità scolastica. Ebbene, la risposta che ci è pervenuta, pur a fronte di tempi ristretti, è stata molto buona e superiore alle nostre attese. Con particolare riferimento al liceo del *made in Italy*, infatti, le istanze sono state

richieste - per nulla scontato, soprattutto se confrontato con simili esperienze del passato. Mi riferisco, ad esempio, al caso del liceo sportivo, introdotto nel 2013 dal Governo Monti, in occasione del quale, nella logica proprio di un avvio graduale di nuovi percorsi e della necessità di un loro monitoraggio nella fase iniziale, vi erano addirittura limiti legislativi che ne contingentavano il numero, prevedendo l'istituzione massima di uno per provincia. Tra le istanze ricevute poi (tranne sei, che sono state escluse per difetto di alcuni requisiti essenziali), tutte le altre hanno ricevuto l'intesa delle Regioni, eccettuato il caso della Campania, che non ha ancora approvato 22 istanze, pur provenienti dalle scuole del proprio territorio. A dispetto di quanto asserito dagli interroganti, le scuole italiane hanno ben compreso la potenzialità di questo percorso, che fornirà alle studentesse e agli studenti la possibilità di approfondire gli scenari sociali, storici, geografici, artistici e culturali dello sviluppo industriale e del tessuto produttivo del nostro Paese, ma anche di proiettarsi nel futuro con una solida formazione di base, soprattutto in campo economico, giuridico e tecnologico. Gli obiettivi formativi e i contenuti qualificanti di tale percorso sono ben scolpiti e precisati nella norma di legge, pur essendo stato delineato al momento il quadro orario del solo primo biennio; ciò è avvenuto anche in occasione della precedente riforma dei professionali fatta nel 2017 dal Governo di centrosinistra. Questa circostanza è stata resa necessaria, come anche in passato, dalla scelta di intervenire con il regolamento attuativo, per individuare in tale sede gli accorgimenti e le compensazioni necessarie a garantire integralmente - sottolineo integralmente, perché è un nostro punto fermo - gli organici dei docenti.

di scuole che hanno aderito a questo nuovo percorso, cioè 120. Va detto che il rispetto, che lei ha ricordato, attiene io credo all'autonomia scolastica, che è stata una riforma importante La domanda era innanzitutto non solo su questo liceo del *made in Italy* e quindi sul fatto che è stato disegnato solo il biennio, su come si farà il triennio, ma soprattutto su come si costruiranno le classi di concorso per gli insegnanti, sulle nuove materie e anche sul rammarico per la scomparsa e la riduzione delle scienze sociali. pensiamo infatti che, tra gli obiettivi formativi di una cittadinanza complessa come quella del nostro tempo, le scienze sociali rivestono un ruolo importante per capire la complessità e per formare le persone alla capacità

Ministro, lei sa che Italia Viva è impegnata in battaglie direi molto complesse, ma al tempo stesso molto giuste, sul tema della sanità. È stato così sulla questione dello *screening* neonatale; a tal proposito, la vogliamo ringraziare per aver accettato la nostra richiesta di istituire lo *screening* neonatale e quindi di firmare il decreto. Ed è così sulla nostra battaglia per il contrasto ai disturbi alimentari. Nel corso della legge di bilancio voi non avete rifinanziato una misura importantissima, che era stata invece portata avanti dal Governo Draghi e che in due diverse annualità, nel 2022 e nel 2023, aveva previsto uno stanziamento di circa 25 milioni di euro. Sono circa 3 milioni le persone che sono attualmente in cura per disturbi alimentari; il dato è quasi triplicato. Si tratta di persone che hanno una media di età di trentacinque anni. C'è un'attenzione specifica, dopo la vicenda della pandemia, perché tutta quella fase nella quale la socialità e la scuola sono state chiuse e ridimensionate ha avuto un effetto importante sui nostri ragazzi. C'è un dato ancor più allarmante: abbiamo pochissime strutture che sono in grado di affrontare questo tipo di disturbo. La metà di tali strutture si trovano al Nord e meno della metà delle strutture sono in grado di ospitare ragazzi di circa anni. Non abbiamo sostanzialmente quasi rete assistenziale al Sud. Anche per questo, Ministro, noi facciamo una battaglia unitaria sul tema della sanità, che non divida il Paese. Purtroppo, infatti, questo genere di disturbo può capitare a chiunque e e avere la consapevolezza di un Paese che non è in grado di affrontare con una rete adeguata questo genere di difficoltà, che per le famiglie può essere devastante e per le persone coinvolte ovviamente può essere letale, è davvero una grave emergenza. per quale motivo questo stanziamento era stato tolto e, visto che ha annunciato a mezzo stampa che ci sarà un ripristino di circa 10 milioni, se invece di fare una misura che duri soltanto un anno, non sia sua intenzione dare stabilità a questo tipo di intervento e renderlo costante nel corso degli anni per attuare una misura preventiva in grado di aiutare le famiglie nel corso del tempo.

A queste misure, dal conferimento del mio mandato, ho sempre rivolto molta attenzione, specie per la grande diffusione di questi disturbi tra i giovani. La legge di bilancio del 2022, come ricordato, nelle more dell'aggiornamento dei LEA, aveva previsto l'istituzione di un fondo, con dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni per l'anno 2023. Per definire la ripartizione complessiva del fondo, nel mese di marzo 2022 è stato istituito un apposito gruppo tecnico-scientifico. I criteri, le linee di intervento per l'utilizzo del fondo e le procedure per la presentazione dei piani di attività biennali da parte delle Regioni e delle Province autonome, elaborate dall'anzidetto gruppo tecnico-scientifico, sono stati oggetto di intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Le risorse sono state quindi ripartite ed entro il 31 ottobre del 2024 le Regioni e Province autonome dovranno trasmettere una relazione e rendicontazione finanziaria. Come previsto, le Regioni e Province autonome hanno presentato al Ministero della salute una relazione intermedia dell'attività svolta nel mese di dicembre scorso. Ad oggi, dalle relazioni intermedie presentate si evince che Regioni e Province autonome hanno impiegato il 59 per cento del finanziamento e speso solo il tre per cento del finanziamento. Ciò premesso, ho comunque contestualmente provveduto, secondo quanto previsto dai commi dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022 nn. 688 e 689, in primo luogo ad adottare 23 giugno 2023, recante la definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale, grazie al quale, dopo molti anni, è possibile dare concretezza al decreto del Presidente per cui ad oggi gli assistiti affetti da anoressia e bulimia possono vedere soddisfatto il loro diritto di usufruire in esenzione delle prestazioni di specialistica ambulatoriali approvate per il monitoraggio del disturbo. L'entrata in vigore del nomenclatore, su unanime richiesta delle Regioni, è riprogrammata al 1° aprile prossimo. Nell'ambito dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, gli assistiti possono accedere a 16 nuove prestazioni di specialistica ambulatoriale. Fermo restando queste prestazioni, nell'ambito della proposta di aggiornamento LEA, la Commissione nazionale per l'aggiornamento LEA e la promozione del Servizio sanitario nazionale ha rilevato l'importanza di introdurre ulteriori nuove 16 prestazioni di assistenza ambulatoriale da concedere in esenzione. Ciò considerato, nelle more della piena operatività del nuovo nomenclatore tariffario e dell'ulteriore aggiornamento dei LEA, atteso per il primo semestre di quest'anno, per garantire ai pazienti affetti da disturbi del comportamento alimentare un'appropriata presa in carico da parte delle strutture regionali, si è in ogni caso deciso, con un emendamento che è stato proposto in sede di conversione al decreto mille proroghe, di mettere a disposizione del fondo straordinario, pur in assenza della completa rendicontazione da parte delle Regioni e di quanto già erogato a loro favore, una cifra pari - come lei ha ricordato - a 10 milioni di euro per il 2024. Resta fermo che con l'entrata in vigore del nuovo nomenclatore tariffario e dell'ulteriore aggiornamento dei LEA sarà garantita finalmente la piena copertura finanziaria in modo strutturale per l'erogazione delle prestazioni a beneficio di tutti i pazienti con disturbi del comportamento alimentare, rendendo di fatto non più necessario qualsivoglia fondo straordinario a carattere temporaneo, come finora sperimentato.

Circa il tema che alcuni degli stanziamenti oggetto di intervento, per esempio, come nel caso specifico, del contrasto ai disturbi alimentari, possono non essere tutti

vorrei dirle che questo Governo interviene sul tema della polemica dei tagli più o meno sempre con la stessa modalità: siccome le Regioni non riescono a spendere bene le risorse, allora il Governo nazionale le taglia. Questo non può essere un criterio, signor Ministro, perché il vostro dovere come Governo è quello di riformare:

impostato e che, a mio modo di vedere, sarebbe stato devastante come messaggio nel Paese, perché aver tagliato anche solo per un giorno quei 10 milioni è un messaggio di grave disattenzione nei confronti di quelle famiglie. Vi siete corretti, l'avete ripristinato, ora l'obiettivo è quello di renderlo strutturale. Avrete in Italia Viva un atteggiamento attento, ma al tempo stesso anche in grado di dire con grande franchezza quando le cose vengono fatte. Per ora avete corretto un errore commesso da voi stessi; avete dato un messaggio sbagliato alle famiglie, ma lo avete parzialmente corretto, quindi avete un'occasione. Al decreto-legge mille proroghe un emendamento proprio di Italia Viva che prevede lo stanziamento di 20 milioni e rende strutturale questo fondo. Approvatelo e avrete la possibilità di dare alle famiglie un messaggio giusto in un momento di grave difficoltà, soprattutto ai nostri ragazzi, perché chiunque può avere un momento di difficoltà, anche dal punto di vista dei disturbi alimentari. L'importante è trovare uno Stato, delle istituzioni, in grado di costituire una rete adeguata per aiutare quelle famiglie e quei ragazzi. È nostro dovere ed è il dovere che noi abbiamo per guardare con fiducia al futuro.

Signor Ministro, lei sa bene che l'Italia è il Paese con la popolazione anziana tra le più longeve al mondo. La popolazione anziana non autosufficiente in Italia è destinata a crescere e questo aumento, insieme al numero delle persone con disabilità, rappresenta una sfida cruciale per il nostro sistema sanitario nazionale. Attualmente solo il 6 per cento delle persone non autosufficienti è ospitato in strutture residenziali; cento delle persone non autosufficienti riceve assistenza dai *caregiver* e per i due terzi del totale la cura è affidata esclusivamente ai familiari, con il supporto solo parziale di strutture semiresidenziali o di servizi di assistenza domiciliare. Signor Ministro, come lei sa, nel marzo 2023 questo Parlamento ha approvato a larga maggioranza una legge che delega il Governo ad attuare diversi decreti attuativi. Era una legge attesa da oltre 8 milioni e mezzo di italiani che hanno nelle loro famiglie persone non autosufficienti o disabili.

la concretezza di queste riforme quali interventi sono previsti nei decreti attuativi in materia di politiche in favore delle persone anziane non autosufficienti e, soprattutto, quali risorse pensate di stanziare, affinché questi interventi possano davvero dare una risposta e un sollievo ai tanti italiani che hanno in casa persone anziane non autosufficienti o persone con disabilità.

agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33, in materia di invecchiamento attivo, promozione dell'inclusione sociale, prevenzione della fragilità, assistenza sociale e sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, politiche per la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a queste persone. Sul provvedimento sarà acquisita l'intesa della Conferenza unificata e trasmessa alle Camere per il prescritto parere. In particolare, il decreto, tra le misure a sostegno della persona anziana, prevede interventi per prevenire la fragilità, promuovere la salute e l'invecchiamento attivo anche nei luoghi di lavoro, favorire l'inclusione sociale e la mobilità. Inoltre, al fine di consentire il mantenimento delle migliori condizioni di vita delle persone anziane presso il proprio domicilio, viene promosso l'impiego di strumenti di sanità preventiva e telemedicina. Per incentivare il dialogo intergenerazionale, sono contemplate iniziative di incontro tra studenti e persone anziane nelle istituzioni scolastiche e nelle università, progetti di servizio civile a favore delle persone anziane, attività fisica, sportiva e benessere psicologico. Parallelamente, vengono previsti il riordino, la semplificazione e il coordinamento delle attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti mediante la valutazione multidimensionale unificata per l'accesso ai servizi sociali e sociosanitari mediante i punti unici di accesso che hanno sede operativa presso le case della comunità. In particolare, si introduce il Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente, individuando i livelli delle prestazioni sociali da erogare per l'assistenza domiciliare sociale integrata con i servizi sanitari. Si prevedono misure per contrastare l'isolamento relazionale, la marginalizzazione delle persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie. Si promuove l'implementazione dei servizi di comunità che operano secondo logiche di rete e di sussidiarietà orizzontale. Laddove emergano fabbisogni di cure e assistenza è prevista la redazione di progetti di assistenza individuale integrati che contiene gli obiettivi di cura, individua gli interventi secondo la durata e l'intensità del bisogno, le figure professionali coinvolte, il *budget* di cura assistenziale ed è sottoposto a monitoraggio periodico. I risultati sono resi disponibili su piattaforme interoperabili. Vi sono inoltre disposizioni volte a garantire l'integrazione degli istituti dell'assistenza domiciliare integrata e del servizio di assistenza domiciliare. Si ribadisce poi il diritto delle persone anziane alla somministrazione di cure palliative e viene introdotta, in via sperimentale, la prestazione universale erogata sotto forma di trasferimento monetario e di servizi alla persona. Vengono definiti gli *standard* formativi e i percorsi di formazione per il personale addetto all'assistenza e al supporto delle persone anziane non autosufficienti, nonché misure volte a sostenere il progressivo miglioramento delle condizioni di vita dei *caregiver* familiari. Per l'attuazione delle suddette iniziative sono messe a disposizione risorse finanziarie pari a circa un miliardo di euro.

di nuovo su altri decreti attuativi relativi ai temi sanitari che interessano gli italiani. Lei ha parlato di misure che rientrano effettivamente in quelli che erano i criteri della legge delega

dalle associazioni firmatarie del patto per un nuovo *welfare* sulla non autosufficienza, che si parla di un fabbisogno di circa 1,306 milioni, di cui 835 milioni della sanità e 471 milioni del sociale.

che il Ministero ha sottoposto al vaglio della Conferenza Stato-Regioni, con i vari obiettivi che si prefigge a tutela della salute dei cittadini italiani e della tenuta del tessuto socioeconomico del nostro Paese. Devo dire che abbiamo molto apprezzato che il documento evidenzi quanto siano importanti i vaccini nel contrasto alla pandemia e il loro spiccato valore solidaristico di tutela delle persone Grazie. a volte per tutelare la salute in un contesto emergenziale sia anche necessario ricorrere alla limitazione delle libertà dei singoli e della collettività per minimizzare i rischi. Altrettanto importante, per noi, è stato poter leggere come il Presidente del Consiglio sia la figura più adatta

alla luce di quanto sopra, io le chiedo quali siano le differenze che presumevamo di vedere marcate tra questo piano strategico e le misure e le misure adottate nell'emergenza pandemica da Covid-19; quali azioni intenda intraprendere per superare le criticità che stanno sollevando le Regioni in merito alle risorse necessarie per realizzare i piani pandemici regionali; in che modo il suo Ministero intenda superare il vincolo dei tetti di spesa per il personale, per ottenere il rafforzamento delle dotazioni organiche per i dipartimenti di prevenzione, per le strutture di livello regionale, per le finalità previste dal piano, tenendo ben presente

senatrice Pirro, avrei voluto parlare di un documento ufficiale e non di bozze. Però, per rispetto delle istituzioni, mi trovo a rispondere a frasi estrapolate da una bozza che è in continua evoluzione. L'obiettivo principale di questo piano strategico è quello di proteggere la salute e la sicurezza della popolazione, garantendo il più possibile l'accesso alle cure mediche durante una improvvisa pandemia. La bozza è in discussione presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. È stata predisposta da un gruppo di lavoro che ha incluso rappresentanti delle regioni dell'Istituto superiore di sanità, Aifa, Agenas, Inail, Dipartimento per la protezione civile, Ispettorato generale della sanità militare, Centro nazionale anti pandemico ed esperti designati. Quindi, è frutto di una lunga ed elaborata discussione, che oggi ci porta a recepire gran parte delle integrazioni, osservazioni e modifiche che sono giunte da parte degli interlocutori. Il documento è ancora in fase di revisione, sia attraverso riunioni con il coordinamento tecnico della Commissione salute delle Regioni, sia attraverso revisioni interne con i Ministeri coinvolti, per adeguare il testo alle osservazioni legittime pervenute. Contrariamente al Panflu, non si limita alla preparazione e alla risposta ad una pandemia da virus influenzale A e B, bensì alla preparazione e risposta a pandemie da eventuali patogeni a trasmissione respiratoria, sia virali che batteriche. Il documento rappresenta uno strumento di pianificazione per la fase interpandemica; uno strumento tecnico a supporto delle decisioni che potranno essere adottate ai diversi livelli amministrativi e legislativi e da diversi attori nelle fasi di allerta e risposta. Voglio evidenziare che è un piano per la gestione emergenziale di patogeni potenzialmente ignoti e che descrive ed elenca strumenti attualmente disponibili di sanità pubblica, che potranno essere applicati in maniera graduata, in rapporto all'entità e alla gravità dell'emergenza. La bozza del piano sottolinea l'importanza della collaborazione tra il Ministero della salute, le autorità locali, le istituzioni sanitarie e le popolazioni per affrontare efficacemente una pandemia. Grande importanza viene data soprattutto alla comunicazione e all'informazione alla popolazione. Elemento cruciale è lo sforzo di sistematizzare e valorizzare le strutture di coordinamento, i sistemi di sorveglianza dei sistemi sanitari. Il piano non si limita a prevedere eventuali scenari epidemiologici e misure di contenimento, ma per la prima volta delinea un potenziale di servizi indispensabili: dipartimenti di prevenzione, l'emergenza-urgenza, ricerca, rete dei laboratori oltre a un'integrazione tra ospedale e territorio. In merito al vincolo dei tetti di spesa sul personale, stiamo lavorando al graduale sblocco e superamento degli stessi. È evidente che, in caso di pandemia, per garantire sicurezza e assistenza alla popolazione, i tetti verranno riparametrati. Stiamo ovviamente procedendo alla quantificazione economica relativa al dettaglio dei costi derivanti dall'implementazione degli interventi descritti, all'illustrazione dei criteri di calcolo per la determinazione dell'importo stimato. Questo è un piano che per la prima volta sarà veramente aggiornato, puntuale, che si attiene scrupolosamente a criteri tecnico scientifici e a direttive internazionali. Questo Governo, rispetto a chi per anni ha fotocopiato un vecchio piano del 2006, prende decisioni con la consapevolezza delle proprie scelte. Mi rincuora leggere i commenti di colleghi autorevoli, che sottolineano come questo sia un piano reale, che rispetta anche la libertà delle popolazioni, fornendo linee guida flessibili, invocando misure restrittive solo come ultima risorsa. È un fatto, non un'opinione, che prima non esisteva un piano pandemico adeguato. Adesso abbiamo e stiamo preparando un documento, che non solo esiste, ma segue tempi e procedure corrette. Questo è un passo in avanti concreto e tangibile verso una gestione più responsabile e preparata alle emergenze sanitarie.

Panflu che nella mia interrogazione non sono presenti, forse ci ha confuso con il Gruppo che segue, quello della Lega, che sì scalpita *(Applausi)* e dà una stoccata a lei, Ministro, sui contenuti del piano. gli attriti di ieri sulle armi all'Ucraina, anche oggi la Lega non vi lesina delle critiche, perché loro hanno qualche problema con le vaccinazioni e le limitazioni delle libertà. Sicuramente non le abbiamo noi. A me preoccupa invece tutelare la salute dei cittadini e questo documento, anche se in bozza, secondo me va nella giusta direzione.

Devo dire che i contenuti di questa bozza - chiamiamola così, anche se sono abbastanza sicura che poi il documento conclusivo non si discosterà molto - mi rincuorano, mi fanno capire e confermano che la Commissione Covid che volete istituire voi della maggioranza è solo una *boutade* e un attacco politico nei confronti di chi vi ha preceduto. *(Applausi)*. Se infatti con questo documento confermate tutte le misure che abbiamo adottato, automaticamente ci state dicendo che quella Commissione è totalmente inutile. Grazie.

non vedono l'ora di scrivere che quello che hanno fatto in passato è tutto giusto. Noi non sappiamo se quello che hanno fatto in passato è tutto giusto perché abbiamo una Commissione che lavorerà apposta per andare a vedere se quello che è stato fatto in passato è tutto giusto. Io credo che si troverà che quello che è stato fatto in passato è molto sbagliato. Pertanto, partendo da questo presupposto, vorremmo sapere dal suo punto di vista, quando e se ci sarà il testo definitivo, dove in particolar modo ci saranno i cambiamenti, e se verranno recepiti all'interno di un piano che sarà un documento politico. Non può essere un documento solo tecnico perché il piano pandemico è quello che poi vincola o quantomeno guida le decisioni future del Governo. Quest'ultimo si è impegnato con i cittadini su tre punti abbastanza importanti: basta restrizioni

L'obiettivo principale del piano strategico 2024-2028 è quello di proteggere la salute e la sicurezza della popolazione, garantendo il più possibile l'accesso alle cure mediche durante una improvvisa pandemia da patogeni potenzialmente non noti. Sottolineo che la bozza del piano pandemico è attualmente in discussione presso la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ed è stata predisposta da un gruppo di lavoro che ha incluso rappresentanti di tutti gli enti interessati e previsti, oltre ad esperti. Essa è frutto di una lunga ed elaborata discussione che ha portato e sta portando a ricomprendere gran parte delle integrazioni, osservazioni e modifiche da parte degli interlocutori. Nello specifico, la bozza è ancora in fase istruttoria, attraverso riunioni con il coordinamento tecnico della commissione salute, area, prevenzione e sanità pubblica, anche al fine di adeguare il testo alle differenti osservazioni espresse dalle Regioni negli ultimi giorni. In relazione alla *governance* delle varie fasi pandemiche, evidenzio che il Ministero della salute, anche su richiesta delle Regioni, sta definendo a livello nazionale regionale ruoli, competenze e tempistiche dei soggetti coinvolti, con il coinvolgimento anche degli altri Ministeri interessati (Ministero dell'istruzione e del merito, Ministero dell'interno, Ministero dei trasporti, Ministero delle infrastrutture, Ministero delle imprese e del Made in Italy, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero del turismo). Certamente in un piano pandemico non è indispensabile citare aspetti giuridici, che esulano dallo scopo dello stesso piano. Sento in ogni caso di dover precisare che, per affrontare un patogeno ignoto con un alto o altissimo tasso di mortalità, potrebbe essere necessario adottare misure restrittive che dovranno però essere emanate solo se strettamente indispensabili, rimanere eventualmente in vigore per il tempo strettamente necessario, essere proporzionali sia alla probabilità sia all'entità dell'evento. Rispetto alle modalità di assunzione delle decisioni in corso di pandemia, qualora non dovesse risultare sufficiente per il governo complessivo della molteplicità di interessi e di settori incisi dall'emergenza sanitaria, la scelta di uno strumento legislativo attraverso il coinvolgimento del Parlamento appare il mezzo più idoneo per garantire l'unità di indirizzo dell'azione di Governo e di bilanciamento dei molteplici interessi pubblici. Ribadisco che il documento è ancora in fase istruttoria. Rispetto infine al tema della discontinuità, appare ultroneo rimarcare che il vecchio piano riguardava la risposta ad un'eventuale pandemia da virus influenzali A e B, mentre l'attuale piano riguarda la risposta ad una pandemia di patogeni respiratori potenzialmente ignoti. In conclusione, vorrei che consideraste questo piano pandemico come una strategia preventiva che ora finalmente abbiamo per la protezione della nostra comunità. È progettato per mobilitare ogni risorsa e azione necessaria in proporzione alla gravità di un'eventuale emergenza, sempre con l'obiettivo supremo di preservare ciò che è più prezioso:

la lunga digressione giuridica che, come può ben immaginare, poco c'entrava e, secondo me, poco era adatta come collocazione, anche perché sembrava una

detto in premessa, magari si volevano autoassolvere. Per il resto, invece, mi fa molto piacere constatare la sua disponibilità al cambiamento del testo. Si ricordi ovviamente nella stesura definitiva i punti che abbiamo preso preso come impegno nei confronti dei nostri cittadini e che sono superiori a qualsiasi considerazione tecnica, pratica o giuridica, perché noi siamo rappresentanti dei cittadini e siamo qui apposta per fare quello che abbiamo promesso loro. *(Applausi)*.

l'impatto di queste attese non è solo un fattore di stress e ansia per i pazienti, ma può anche comportare un aggravamento delle condizioni di salute e un aumento dei costi per il sistema sanitario; il malgoverno del passato ha lasciato un'eredità di inefficienze, che necessitano di un intervento deciso e di una visione strategica capace di trasformare in profondità il nostro sistema di assistenza sanitaria; In questo scenario la nomina di lei, signor Ministro, alla guida del Dicastero della salute è stata accolta con fiducia e speranza. La sua affermata carriera nel campo medico e la capacità di visione strategica che ella sta dimostrando sono elementi che nutrono la convinzione di una svolta imminente e positiva, a tutela e rilancio del Servizio sanitario nazionale. Fatta questa premessa, le chiediamo di sapere quali azioni concrete ella, signor Ministro, intende intraprendere per affrontare la grave problematica delle liste d'attesa per le prestazioni sanitarie, anche in considerazione dell'aumento di risorse stanziate a favore del fondo sanitario nazionale.

senatrici e senatori interroganti, perché mi offrono la possibilità di illustrare le iniziative che il Ministero sta mettendo in campo per consentire, con un compiuto riordino della rete territoriale, il recupero dei tempi delle liste d'attesa, garantendo una prima risposta efficace sul territorio. In proposito, anche dall'analisi del rapporto civico sulla salute 2023 di Cittadinanzattiva, emerge che, terminata l'emergenza pandemica, i cittadini si trovano a fare i conti più di prima con le conseguenze di scelte improvvide, che durano da decenni; scelte che, come ho già avuto modo di evidenziare, hanno ottenuto un solo e unico effetto: un sistema sanitario nazionale ingolfato, senza interventi strutturali. Le liste d'attesa non sono altro che il sintomo di un sistema da ripensare. da ripensare l'architettura complessiva dell'offerta sanitaria, con il potenziamento della medicina territoriale. Sono allo studio proposte concrete per l'implementazione del sistema disegnato dal decreto interministeriale n. 77 del 2022, con sistemi di telemedicina e di supporto specialistico-diagnostico integrato, per soddisfare al meglio i bisogni degli assistiti,

e Province autonome nell'attuazione di quanto disposto, il Ministero ha diramato uno specifico atto di indirizzo per dare indicazioni specifiche sulle attività di recupero delle prestazioni ambulatoriali, *screening* e ricovero ospedaliero, per ridurre le liste d'attesa, garantendo nel contempo il prosieguo delle attività di monitoraggio e supporto fornito da Agenas. Sempre con l'obiettivo di ridurre le liste d'attesa, rappresento che, con la legge n. 213 del 2023, viene previsto un rifinanziamento dei piani operativi per l'abbattimento delle liste d'attesa, per cui le Regioni potranno utilizzare una quota non superiore allo 0,4 per cento del livello di finanziamento indistinto, per un ammontare, per l'anno 2024, di 520 milioni di euro. A ciò si aggiunge l'aumento della tariffa oraria per le prestazioni aggiuntive dei medici (100 euro) e del personale sanitario (60 euro), nonché l'autorizzazione alla spesa di 200 milioni di euro per il personale medico nel 2024 e di 80 milioni di euro per il personale sanitario del comparto sanità. Per garantire la completa attuazione dei piani operativi per il recupero delle liste d'attesa, le Regioni e Province autonome potranno avvalersi anche del coinvolgimento di strutture private accreditate. Tra le iniziative intraprese, voglio ricordare che il Ministero della salute ha istituito il tavolo tecnico per l'elaborazione e l'operatività del Piano nazionale di governo delle liste d'attesa 2024-2026, a cui è stato attribuito il compito di portare a termine la nuova pianificazione nazionale in materia e i nuovi meccanismi di monitoraggio e controllo. Fatemi sottolineare che, in conclusione, la situazione delle liste d'attesa dimostra che i fondi servono, ma ciò che soprattutto serve è saperli spendere bene. Questa però è la prima volta che abbiamo un piano che, oltre a stanziare fondi *ad hoc*, si impegna a realizzare una riorganizzazione strutturale. Fatemi aggiungere una nota polemica: la nostra attenzione è unicamente dedicata a soluzioni permanenti e non emergenziali. Al gettonismo indegno ed esageratamente oneroso vogliamo recuperare ed attuare definitivamente il modello auspicato quarantacinque quando nacque il nostro Servizio sanitario nazionale, ovvero qualità delle prestazioni, con una gestione sostenibile dei fondi a disposizione. La sfida è anche nelle mani delle Regioni, ma il Ministero non mancherà di supportare le buone pratiche e di intervenire con ogni mezzo nelle realtà incapaci di garantire almeno i livelli essenziali di assistenza.

a concreta difesa e rilancio di un Servizio sanitario nazionale pubblico e universalistico. Com'è stato ricordato più volte, con la legge di bilancio 2024 in tre anni sono stati destinati 11,2 miliardi di euro in più al Fondo sanitario, che rappresenta il più alto investimento mai fatto. Le misure che lei ci ha illustrato per ridurre la piaga delle liste d'attesa rappresentano certamente un tassello importante di una più ampia strategia di rilancio del nostro sistema sanitario pubblico, così come della massima importanza riteniamo l'attenzione che il Governo e lei, signor Ministro, sta dimostrando nel valorizzare il personale sanitario, con misure che erano attese da anni. Mi riferisco allo stanziamento di 2,4 miliardi di euro per il rinnovo contrattuale, all'incremento degli straordinari degli operatori del pronto soccorso, alle misure a difesa degli stessi dal gravissimo fenomeno delle aggressioni e a molto altro ancora. Difficile sostenere che in poco più di un anno si potesse fare di più. Non riconoscerlo e attribuire a questo Governo criticità che originano da oltre dieci anni di definanziamento e gravi carenze di programmazione è a dir poco ingeneroso. Allora, signor Ministro, nel ringraziarla, la incoraggiamo a proseguire nella sua complessa opera di tutela e rilancio del nostro Servizio sanitario nazionale.